le senatrici Puppato e Bignami, unitamente ad altri senatori, richiamano l'attenzione del Ministro dell'interno sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati, chiedendo di adottare incisive misure, anche di natura normativa, per assicurare più elevati livelli di accoglienza e un maggior sostegno finanziario ai Comuni impegnati in prima linea. Le problematiche legate all'accoglienza di tali minori sono da tempo all'attenzione del Ministero dell'interno, anche in ragione del fatto che, nell'ambito degli ingenti flussi migratori che stanno interessando il territorio nazionale, si registra un numero crescente di arrivi di questa categoria di soggetti vulnerabili. I dati relativi ai minori in questione, tenuti aggiornati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mostrano chiaramente che negli ultimi quattro anni l'afflusso dei minori non accompagnati è sostanzialmente raddoppiato, essendosi passati dalle 5.821 unità presenti in Italia nel 2012 alle 11.921 dell'anno scorso. L'*escalation* del fenomeno ha reso pressante l'esigenza di assicurare un adeguato supporto dello Stato ai Comuni ai quali spettano - come è noto - l'assistenza e la rappresentanza legale dei minori fuori famiglia. In tale direzione vi è stato un radicale ripensamento della *governance* del sistema nazionale di accoglienza, con una contestuale forte assunzione di responsabilità del Ministero dell'interno. Il nuovo sistema ha avuto origine con il piano operativo nazionale per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 luglio 2014, la cui portata innovativa risiede nel fatto che, ferma restando la prioritaria competenza dei Comuni, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati vede il coinvolgimento a regime dei tre livelli di Governo del Paese: lo Stato, le Regioni e gli stessi Comuni che hanno deciso di condividere i relativi oneri in maniera proporzionale e secondo parametri predefiniti sul territorio. Un ulteriore tratto distintivo del nuovo sistema sta nell'averlo strutturato - proprio nel senso auspicato dalla senatrice Bignami in modo che l'accoglienza dei migranti fuoriesca dalla logica emergenziale praticata in passato, anche attraverso il ricorso a strumenti propri della Protezione civile, per acquisire la connotazione di attività ordinaria, strutturale e programmabile. Le previsioni del piano nazionale hanno poi trovato suggello e copertura in due interventi legislativi. Mi riferisco, innanzitutto, alla legge di stabilità 2015 che - come riportato nell'interrogazione della senatrice Puppato ha trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno il fondo destinato a sostenere finanziariamente i Comuni che erogano i servizi di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati. Si è trattato di un'importante misura di razionalizzazione, in quanto, superando precedenti frammentazioni, ha consentito di concentrare in un unico Dicastero gli interventi di competenza statale nel settore dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Si ritiene che questo accorpamento abbia rappresentato un vero passo in avanti, tenuto conto del consolidato rapporto di collaborazione che il Viminale ha tradizionalmente costruito con gli enti locali, i quali sono gli effettivi terminali sul territorio di questo delicatissimo problema. La stessa legge di stabilità 2015 ha previsto, d'altro canto, la possibilità di ospitare nelle strutture dello SPRAR, gestite come noto dagli enti locali con la regia unitaria e il preponderante sostegno finanziario del Ministero dell'interno, i minori stranieri non accompagnati non richiedenti protezione internazionale. Si è trattato anche in questo caso di un'innovazione di non poco conto, atteso che il sistema SPRAR è destinato tradizionalmente all'accoglienza dei soli richiedenti asilo e rifugiati. Più di recente, è intervenuto il decreto legislativo n. 142 del 2015 che, attraverso varie disposizioni di chiarificazione e chiusura del sistema, ne ha disegnato i contorni con maggiore precisione. Il dispositivo normativo prevede una fase di prima accoglienza del minore in strutture ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'interno. La permanenza in tali centri è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non è superiore a novanta giorni. Il minore è successivamente ospitato nelle strutture di seconda accoglienza del sistema SPRAR gestite - come detto - dai Comuni secondo un modello condiviso con il Ministero dell'interno, che valorizza l'ospitalità diffusa e mira all'integrazione. Qualora tali strutture siano temporaneamente indisponibili, gli enti locali provvedono comunque a ospitare il minore attraverso i propri servizi di assistenza, secondo i criteri di ripartizione su base regionale individuati, previa intesa con la Conferenza unificata, dal tavolo nazionale di coordinamento operante presso l'Amministrazione dell'interno, nel quale il mondo delle autonomie locali è comunque ampiamente rappresentato. In tal caso, i Comuni possono fare richiesta di accedere, nei limiti delle risorse disponibili, al già citato fondo del Ministero dell'interno. Segnalo al riguardo - e con questo rispondo a un altro dei quesiti delle senatrici interroganti - che il fondo ha ricevuto per l'anno in corso una dotazione finanziaria importante: si tratta di 170 milioni di euro (cioè quasi il doppio dei 90 milioni assegnati per il 2015) che si ritiene possano contribuire a elevare in maniera significativa gli *standard* qualitativi e quantitativi dell'accoglienza. Le somme relative al 2015 pari - come appena detto - a 90 milioni di euro, sono state già assegnate e pagate ai Comuni richiedenti per il 92 per cento dell'importo complessivamente stanziato. Per l'anno in corso sono già iniziati i pagamenti relativi al primo trimestre. È evidente che la consistenza del fondo può essere ulteriormente incrementata e, anzi, è auspicabile che ciò avvenga, ma occorre a tal fine un mirato intervento legislativo che dovrà farsi carico di reperire la necessaria copertura finanziaria. Questi sono gli aspetti salienti del nuovo sistema di accoglienza dei minori non accompagnati. È stato importante riepilogare l'intero modello organizzativo, pur nella consapevolezza di fornire notizie in parte già conosciute, per evidenziare come esso realizzi un significativo sostegno dello Stato ai Stato ai Comuni. Si tratta, comunque, di un sistema ancora in fase di costruzione e che, quindi, non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Per quanto riguarda la prima accoglienza, l'Autorità responsabile del fondo europeo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione ha pubblicato, lo scorso 22 aprile con scadenza ieri, 22 giugno, il bando il bando pubblico necessario all'allestimento dei primi mille posti ad alta specializzazione. Nelle more, per fronteggiare le esigenze più pressanti, abbiamo attivato strutture temporanee di accoglienza per oltre 700 minori al giorno nel 2015 e per 614 minori al giorno fino al prossimo 22 agosto, utilizzando anche in questo caso risorse del fondo europeo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione. Per quanto riguarda la seconda accoglienza, informo che la rete SPRAR, già dotata di circa 2.000 posti dedicati ai minori non accompagnati, sarà potenziata a breve con ulteriori 2.000 posti, per i quali si è già provveduto a diramare l'avviso pubblico. Voglio evidenziare che con tale bando, per la prima volta, la compartecipazione dei Comuni alle spese da sostenere per la creazione dei posti

Ritengo di poter dire che il Governo sta dedicando la dovuta attenzione ai minori non accompagnati e che l'Amministrazione dell'interno, in particolare, si sta adoperando per assicurare loro un'accoglienza in linea con le politiche europee di settore e rispettosa dei principi sanciti dalle convenzioni internazionali siglate dall'Italia. Tutto ciò in stretto raccordo con l'ANCI e gli altri organi rappresentativi delle autonomie locali, con i quali vi è, per espressa disposizione di legge, una costante interlocuzione e condivisione delle scelte e delle strategie da mettere in campo sia in sede di Conferenza unificata che nell'ambito del citato tavolo nazionale di coordinamento presso il Viminale e dei tavoli regionali operanti presso le prefetture dei capoluoghi di Regione. Siamo consapevoli che, nella gestione di un fenomeno così complesso, possono verificarsi delle criticità. Ma vi è l'impegno da parte nostra a fronteggiarle, impiegando, anche in futuro, ogni nostra risorsa per l'effettivo rispetto dei diritti dei minori stranieri non accompagnati, in adesione ai principi universali di tutela della persona, che sono alla base della nostra civiltà giuridica.

all'incremento del fondo dei 170 milioni cui lei accennava, Vice Ministro, associato ancora al fatto che è già stata predisposta una serie di autorizzazioni per 2.000 posti (e ulteriori 2.000 posti) per minori,

di monitorare questo importantissimo fenomeno, di gestirlo adeguatamente e soprattutto di tutelare le economie di quei Comuni che in maniera così sensibile ritengono di ospitare questi minori. Quindi, mi ritengo pienamente soddisfatta della risposta e ringrazio moltissimo il Ministero, auspicando, signor

il Parlamento, in particolare il Senato in cui sediamo oggi, credo dovrà farsi carico, laddove serva, di implementare adeguatamente i *plafond* e le normative disponibili per lo specifico settore del mantenimento dei minori non accompagnati.

il dato certo che i non rintracciabili sono 6.135: quindi raddoppiano le entrate e raddoppiano i non rintracciabili. Vorrei porre l'attenzione su questo numero,

alimentano il male e tutto ciò che concerne l'ombra oscura di cui non si parla mai. I 6.135 non hanno davanti un grande destino e lo sappiamo. Sono ragazzini che vengono utilizzati dal malaffare:

chiede che l'Opera di Santa Maria del Fiore faccia chiarezza sull'effettiva destinazione dei fondi raccolti dall'Unicoop di Firenze per finanziare il restauro del Battistero di San Giovanni. Premetto che l'Opera di Santa Maria del Fiore, in quanto fabbriceria, è soggetta al regime di controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 33 del 1987, in base al quale il Presidente dell'ente è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il bilancio di previsione dell'anno successivo e, entro il 31 marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'anno precedente. I due documenti contabili, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio di amministrazione della fabbriceria. sentito il vescovo diocesano, qualora siano accertate gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero l'impossibilità per la fabbriceria di continuare a funzionare, può sospenderla, ove ricorrano motivi di urgente necessità, affidandone la provvisoria gestione a un suo commissario. In ogni caso, egli riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il vescovo diocesano e udito il Consiglio di Stato, può sciogliere l'ente e nominare un commissario straordinario. Ciò chiarito in linea generale, evidenzio che l'Opera del Duomo ha regolarmente depositato presso la prefettura di Firenze i conti consuntivi e i bilanci di previsione. Secondo quanto riferito dal prefetto, i consuntivi relativi agli anni 2014 e 2015 hanno registrato un utile di esercizio rispettivamente di 3 e di 2,6 milioni di euro circa, mentre l'utile stimato per il 2016 ammonta a circa 1,5 milioni di euro. La conformità dei predetti consuntivi alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione è stata regolarmente certificata dalla società di revisione incaricata. Queste sono le risultanze dei controlli del prefetto, che evidenziano il rispetto degli obblighi contabili e sembrano confermare una solida situazione finanziaria dell'Opera. Riguardo alle specifiche richieste degli interroganti sull'utilizzo dei fondi raccolti da Unicoop, l'Opera ha comunicato che nell'ultimo triennio si è reso necessario uno straordinario intervento manutentivo riguardante il battistero, le facciate dei tre grandi palazzi prospicienti il lato sud del Duomo, le rovine dell'antica cattedrale di Santa Reparata e il museo, con il restauro di trecento opere d'arte; interventi del valore totale di oltre 40 milioni di euro. I relativi impegni finanziari sono stati affrontati utilizzando, in parte, le risorse accantonate negli anni precedenti e, in parte, gli utili gestionali conseguiti anche grazie a una complessiva opera di controllo dei costi e ad alcune operazioni di natura commerciale e di *marketing*, che hanno consentito di passare dai 10,4 milioni di euro d'incasso nel 2010 (anno di subentro dell'attuale consiglio di amministrazione) ai 16,6 milioni di euro d'incasso nel 2015, così da raggiungere nel periodo di riferimento utili complessivi pari a circa 14,5 milioni di euro. Nel contempo, l'Opera ha proceduto a una riorganizzazione interna che ne ha accresciuto l'efficienza operativa, anche attraverso l'introduzione del controllo di gestione e di criteri di imprenditorialità e l'assunzione di 15 importanti figure professionali di età inferiore a quarant'anni. Per sostenere finanziariamente il complesso delle operazioni programmate, l'Opera ha cercato di far ricorso anche alle sponsorizzazioni private, proponendo a oltre 30 grandi imprese fiorentine di associare il proprio nome ai lavori di restauro. Anche a causa di impedimenti e vincoli previsti dal regolamento comunale sulla pubblicità, l'iniziativa non ha trovato adesioni, ad eccezione di un'unica offerta di contributo di circa 60.000 euro. In questo contesto, si colloca la raccolta di fondi promossa da Unicoop tra i propri soci, che ha fruttato complessivamente circa 200.000 euro - precisamente 201.680 euro 201.680 euro - tutti versati nelle casse dell'Opera per concorrere ai costi di restauro del Battistero, ammontanti complessivamente a 1 milione e 970.000 euro. I fondi Unicoop hanno coperto, quindi, poco più del 10 per cento dei costi sostenuti; un altro 6 per cento circa è stato assicurato con il contributo di altri donatori, mentre il rimanente 84 per cento è stato erogato direttamente dall'Opera con risorse proprie. L'Opera ha tenuto a precisare, da un lato, che l'importo totale dei lavori - pari come detto a poco meno di 2 milioni di euro - è stato regolarmente versato alle imprese che li hanno eseguiti sotto il controllo della soprintendenza; dall'altro, che la documentazione specifica sull'utilizzo delle somme raccolte da Unicoop non è stata fornita a Unicoop medesima in maniera approssimativa, bensì utilizzando lo schema di rendicontazione che viene richiesto dal fisco degli Stati Uniti per le donazioni effettuate da imprese americane che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali. L'Opera ha aggiunto che nessuna risorsa pubblica è mai entrata nelle proprie casse. Quanto al 2015, i proventi sono derivati: per l'82 per cento dalla vendita dei biglietti di ingresso ai monumenti; per il 13 per cento dallo sfruttamento commerciale del patrimonio immobiliare e finanziario; per cento da donazioni prevalentemente internazionali. All'interno di tale voce, la donazione Unicoop ha rappresentato solo l'1,2 Quanto all'asserita maxi buonuscita ai due direttori generali succedutisi negli ultimi anni, sempre l'Opera ha informato che, per corrispondere l'emolumento, non sono state utilizzate le somme raccolte né da Unicoop né da altri donatori, ma unicamente le risorse provenienti dalla propria attività istituzionale di organismo privato e non sovvenzionato da alcun contributo pubblico. La buonuscita ha riguardato due dirigenti apicali e ha compreso sia l'indennità di mancato preavviso che le indennità supplementari, in linea con i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e con quanto sancito in sede di conciliazione davanti alle rispettive rappresentanze sindacali. Nella quantificazione dell'importo si è tenuto conto anche degli importanti risultati raggiunti dai professionisti in termini di efficienza e organizzazione dell'ente. Infine, con riferimento agli eventuali aspetti penali della vicenda, il Ministero della giustizia ha comunicato che la procura della Repubblica di Firenze ha delegato alla Guardia di finanza gli accertamenti preliminari tesi a stabilire la sussistenza o meno di reati. Gli accertamenti sono ancora in corso.

prendiamo atto che sono state riportate con dovizia di particolari, della qual cosa la ringrazio.

pongono all'attenzione del Governo il caso della Lande Srl, società avente sede a Napoli, affidataria di appalti pubblici in diverse zone del Paese e con diverse stazioni appaltanti, e coinvolta, attraverso uno dei titolari, in vicende giudiziarie di natura penale. In particolare, la senatrice Capacchione lamenta che la società continui a intrattenere rapporti contrattuali con varie amministrazioni pubbliche in assenza della prescritta certificazione antimafia e chiede al riguardo di conoscere i motivi che impedirebbero al prefetto di Napoli di assumere le determinazioni di competenza sul rilascio della predetta certificazione o, ricorrendone i presupposti, sull'applicazione dell'interdittiva antimafia. antimafia. Il tema evidenziato è particolarmente seguito in Parlamento, tant'è che su di esso sono stati presentati, nelle scorse settimane, diversi atti di sindacato ispettivo, uno dei quali discusso dallo stesso Ministro dell'interno in sede di *question time* in Aula alla Camera nello scorso mese di maggio. Rispetto a quanto riferito dal Ministro in quell'occasione, è intervenuta - com'è noto - una novità di rilievo proprio nel senso auspicato dai senatori interroganti. Riepiloghiamo le questioni. I rapporti contrattuali della società Lande con le diverse stazioni appaltanti sono stati instaurati in presenza di informative di carattere liberatorio rilasciate dalla prefettura di Napoli fino al 2013. Tali informative - com'è noto - sono suscettibili di successivi aggiornamenti, in relazione a fatti nuovi o anche pregressi che disvelino una compromissione di tipo mafioso dell'operatore economico. Naturalmente in questo caso il codice antimafia prevede l'immediato recesso dell'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente caducazione del contratto, nonché l'estromissione dell'impresa da ogni rapporto in essere con qualsiasi amministrazione pubblica. Avvalendosi delle facoltà di legge, nel 2014 la prefettura di Napoli ha avviato una nuova istruttoria, volta a verificare l'eventuale sussistenza di elementi di infiltrazione o condizionamento della criminalità organizzata a carico della società in questione. I motivi che hanno portato a esercitare una particolare attenzione sulla Lande sono riconducibili a procedimenti penali in cui viene avanzata l'ipotesi accusatoria secondo la quale vi sarebbe stata una strumentalità dell'impresa rispetto alla criminalità casalese. In effetti, il precedente amministratore unico e direttore tecnico della Lande, coinvolto in un procedimento per reati vari, tra i quali quello di turbativa d'asta e turbata libertà di scelta del contraente, è stato raggiunto da una misura cautelare, eseguita tuttavia dopo le sue dimissioni dalle cariche societarie. Preciso che l'attività della prefettura non si è limitata a una disamina della documentazione inerente all'impresa, cioè alla sua compagine societaria e tecnica, ma ha comportato anche l'esecuzione di ispezioni e accessi presso le sede della stessa società e nelle diverse aree di cantiere. Nel caso di specie, vi hanno provveduto sia il gruppo investigativo antimafia, sia lo specifico nucleo interforze preposto alle verifiche *in situ*, secondo la metodologia di controllo antimafia messa a punto per le grandi opere e poi estesa anche agli appalti ordinari. Le verifiche si sono rivelate particolarmente complesse, anche in considerazione del mutato assetto proprietario, che ha visto la trasformazione da società a responsabilità limitata a società per azioni e che si connota ora per la presenza di un soggetto detentore di quote azionarie in qualità di *trust*. Nel frattempo, non è stata presa alcuna decisione neanche in merito alla richiesta avanzata dalla Lande di iscrizione nelle *white list* tenute dalla stessa prefettura di Napoli. È noto, infatti, che solo un esito completamente liberatorio può comportare l'iscrizione negli elenchi prefettizi relativi a particolari settori a rischio, istituiti in ogni prefettura in attuazione della cosiddetta legge Severino del 2012. Gli accertamenti disposti dalla prefettura si sono conclusi con l'adozione, il 3 giugno scorso, di un'interdittiva antimafia nei confronti della Lande. Il provvedimento è stato immediatamente trasmesso alle grandi stazioni appaltanti per l'assunzione dei provvedimenti caducatori ed estromissivi di competenza. Soggiungo che la prefettura di Napoli, in riscontro alla richiesta formulata dall'Autorità nazionale anticorruzione, ha dato avvio al procedimento per l'adozione delle misure gestionali straordinarie e temporanee di cui all'articolo 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; ciò anche in considerazione del rilevante numero di rapporti contrattuali che la società Lande intrattiene con le pubbliche amministrazioni e delle correlate esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali. La sussistenza delle condizioni per l'adozione delle suddette misure straordinarie sarà valutata in un'apposita conferenza di servizi, che è in preparazione e per la quale la prefettura, già la settimana scorsa, ha richiesto alle stazioni appaltanti elementi informativi in ordine ai rapporti contrattuali in corso. Per completezza, informo che, a seguito dell'interdittiva antimafia, la prefettura sta completando il procedimento per il rigetto dell'istanza di iscrizione della Lande nelle *white list*. ringrazio il Vice Ministro per la risposta all'interrogazione e devo dire che non mi sento di esprimere un giudizio, né di soddisfazione né di insoddisfazione, perché mi sembra di capire che la ricostruzione fatta dalle prefetture, in particolare da quella di Napoli, sia durata nove mesi. Pertanto, quando parliamo di controlli per evitare le infiltrazioni, un tempo così lungo

la cui prima firmataria è la collega Capacchione, che ringrazio anche per la qualità dell'esposizione, si basa soprattutto su un problema che ci poniamo come legislatori, signor Vice Ministro, e lo dico soprattutto conoscendo la sua sensibilità, essendo stato amministratore locale. C'è un tema: i controlli preventivi. Non si può immaginare di affidare un appalto a una società che non è iscritta nelle *white list* o che comunque ha presentato un'istanza di reiscrizione, visto che probabilmente non lo era al momento dell'appalto.

Tutti questi artifizi dal punto di vista contrattuale e anche giuridico di fatto vanificano lo sforzo che viene fatto dai legislatori, dai Ministeri e dalle Forze dell'ordine per evitare l'infiltrazione nei Comuni attraverso gli appalti pubblici. Tra le altre cose, c'è un tema che probabilmente ci dobbiamo porre come legislatori, quello cioè della circolarità delle informazioni date da prefetti ad altri prefetti. Se la società Lande ha 28 appalti in Italia (e parliamo di grandi appalti), non è immaginabile che una interdittiva antimafia, emessa dopo nove mesi dal momento della richiesta da parte della prefettura territorialmente competente, nel caso quella di Napoli, debba poi avere un percorso ulteriormente dilatato nei tempi per le altre prefetture. Penso - per esempio - al prefetto di Alessandria,

e il 30 dicembre 2015 ha liquidato uno stato di avanzamento dei lavori, cioè il giorno dopo; mi chiedo quindi come era possibile avere le informazioni in Tra le altre cose, il giorno dopo è stato liquidato uno stato di avanzamento dei lavori (come scritto anche nell'interrogazione presentata da me insieme alla senatrice Capacchione e altri colleghi),

Nel frattempo, nel mentre è arrivata questa interdittiva antimafia, la ditta Lande è stata ampiamente pagata per stato di avanzamento dei lavori dal Comune di Portici e - presumo - anche da altre stazioni appaltanti. appaltanti. Da *ex* amministratore mi chiedo quale sarà il percorso che dovranno fare le stazioni appaltanti per farsi restituire i soldi che sono stati pagati alla società Lande, che non poteva contrarre con la pubblica amministrazione.

che garantisca una circolarità delle notizie. Nella fattispecie, non è possibile che l'interdittiva antimafia rilasciata dalla prefettura di Napoli nei confronti della società Lande abbia bisogno di un altro mese di tempo per essere recepita da altre prefetture. L'interdittiva antimafia è unica e vige su tutto il territorio nazionale e, nel momento in cui è emessa dalla prefettura territorialmente competente, obbliga tutte le altre prefetture e tutte le stazioni appaltanti a recepirla immediatamente. Probabilmente va valutato, anche in sede legislativa,

Nello stesso frangente i legali della ditta mi scrivevano per intimarmi di non parlare male dell'azienda perché ne andava del suo buon nome e, infatti, vediamo quali sono stati i risultati. risultati. Come diceva il collega Cuomo, è grave che si impieghi così tanto tempo a intervenire in situazioni di questo genere, soprattutto per aziende che

Detto questo, auspico che ci siano degli strumenti più celeri per definire situazioni di questo tipo anche perché, nel momento in cui si parla di lavori pubblici e di pubblica amministrazione, i soldi sono dei cittadini e sarebbe meglio

la Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova SpA è concessionaria delle tratte autostradali A4 Brescia-Padova, A31 Agugliaro-Piovene Rocchette e A31 Interconnessione con la strada statale 434-S.Margherita d'Adige, in forza della convenzione unica sottoscritta con l'ANAS il 9 luglio 2007, approvata con legge n. 101 del 2008 e divenuta efficace nel mese di novembre 2009 a seguito dell'archiviazione della procedura di infrazione avviata dall'Unione europea, che ha tra l'altro fissato il termine della scadenza contrattuale rideterminandolo al 2026. Infatti, all'articolo 4, comma 1, della suddetta convenzione è stabilito che la scadenza della concessione è fissata al 31 dicembre 2026, in funzione della realizzazione della Valdastico Nord. Veniva anche stabilito che, qualora il progetto definitivo della Valdastico Nord non fosse stato approvato entro il 30 giugno 2013, sarebbero stati conseguentemente definiti tra le parti gli effetti sul piano economico finanziario (PEF) e sulla convenzione. Tale termine del 30 giugno 2013 è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2015, in accordo con i competenti uffici della Commissione europea. In merito al predetto progetto della Valdastico, il primo lotto (in territorio Veneto) è stato già approvato con delibera del CIPE n. 21 del 2013. In data 6 agosto 2015 il CIPE ha altresì preso atto dell'accordo intervenuto tra il Governo italiano e la Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto in ordine all'*iter* di definizione dell'intesa sulla realizzazione del collegamento autostradale Valdastico Nord, secondo lotto di completamento, tra il casello di Valle dell'Astico e la congiunzione con l'autostrada A22 del Brennero. L'accordo ha previsto la costituzione di un comitato paritetico fra lo Stato, la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento. Il comitato paritetico ha concluso i propri lavori il 9 febbraio 2016, confermando la presenza delle condizioni previste e individuando come scenario migliore la realizzazione di un corridoio d'interconnessione infrastrutturale tra la Valdastico, la Valsugana e la Valle dell'Adige. Al fine di recepire le decisioni del comitato paritetico in relazione alla realizzazione del collegamento autostradale Valdastico Nord, il 14 marzo 2016 la società ha trasmesso una versione aggiornata del piano economico finanziario che, successivamente istruita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata presentata lo scorso 17 maggio al CIPE unitamente alla documentazione di riferimento e contestualmente alla presentazione del documento conclusivo del predetto comitato, al fine della successiva approvazione necessaria per avviare le procedure progettuali della tratta Valdastico Nord secondo lotto, quelle di realizzazione del 1° lotto già approvato e tutte le altre attività necessarie per la realizzazione delle altre opere. Dunque, come ha già avuto modo di riferire in quest'Aula il ministro Delrio la scorsa settimana, in sede di *question time,* per la società Brescia-Padova la concessione non è stata prorogata, bensì è in essere fino al 2026: non si è quindi in presenza di una proroga alla concessione scaduta, ma di attuazione di quanto espressamente previsto nella convenzione vigente. Si ricorda, infine, che della procedura descritta, il ministro Delrio ha dato specifica informazione al Commissario europeo della Direzione generale mercato interno, industria, imprenditoria e piccole e medie imprese, Elzbieta Bienkowska, nonché alla Direzione stessa. in merito alle motivazioni della proroga della concessione dell'autostrada A22, riprendo integralmente quanto ho già avuto modo di riferire poc'anzi al senatore Malan: il 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il protocollo di intesa per l'applicazione del modello di gestione di cui all'articolo 17 della direttiva europea n. 23 del 2014, che prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di affidare direttamente una concessione, qualora vengano rispettati i requisiti ivi previsti. Pertanto, con la sottoscrizione di tale protocollo, non è stata autorizzata alcuna proroga alla concessione. A conclusione della procedura di cui all'articolo 17 secondo quanto previsto dal protocollo, dovrà essere stipulato con la società concessionaria un atto convenzionale, che fissi la durata della concessione, il programma degli investimenti e le modalità di finanziamento.

io chiedo, per l'appunto dal settembre del 2015, di sapere chi ha firmato quelle proroghe senza le quali la società concessionaria sarebbe inadempiente. Nel testo che il Sottosegretario ci ha letto egli dice «è stata prorogata». Il mio professore di storiografia diceva che quando si parla di storia non bisogna usare il verbo passivo perché altrimenti non si capisce chi fa. «È stata»: io da due anni chiedo di sapere chi è il signore o la signora che ha apposto la sua firma a questa proroga. A quanto pare è un problema, perché neanche oggi è stato possibile saperlo. Faccio presente di avere anche fatto un accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241 del 1990. Il mese previsto dalla legge è scaduto senza aver avuto nessuna risposta; ho fatto pertanto ricorso alla commissione per l'accesso. La commissione per l'accesso ha esaurito i suoi trenta giorni sabato scorso ma io ancora non ho notizie. Non so se devo appellarmi a qualche entità superiore. Per quanto riguarda la sostanza, apprendo, ringraziando a tal riguardo il Sottosegretario, di una serie di atti intervenuti e di cui sarebbe stato anche normale

chiaro e avere idea di quali siano questi atti e in che modo è stata modificata questa convenzione. In pratica, nel 2007 è stata data in concessione per ulteriori venti anni, fino al 2026 (ma l'intenzione originaria era quella di fissare una scadenza più lontana), questa importantissima autostrada, che incassa oltre 300 milioni all'anno, alla società che la gestiva già da quasi quarant'anni, se non di più. Questo in ragione del fatto che la suddetta società completasse questa struttura con l'autostrada Valdastico Nord: non con qualunque opera che si chiamasse Valdastico Nord, ma con questa autostrada. Dalle notizie che leggiamo sui giornali, questa autostrada non sarà tale, ma un collegamento o un allargamento dell'attuale statale; sarà qualcosa altro. Non si vede, a questo punto, perché quella convenzione del 2007, che è stata oggetto di attenzione (anzi, vi sono stati dei ritardi perché ci sono state delle eccezioni dell'Unione europea),

E non mi risulta che su questa autostrada si siano ridotte le tariffe. Su questa autostrada le tariffe sono aumentate, negli ultimi dieci anni, del doppio dell'inflazione. Qual era la ragione di tale aumento? Fare le nuove infrastrutture. Ma non sono state fatte, né si faranno. Se ne farà una molto meno cara. Purtroppo siamo siamo ancora nella solita ottica. Faccio notare che, al di là delle considerazioni che si possono fare, gli ultimi dieci anni di questa concessione (cioè dall'anno scorso,

il Ministero o la commissione per l'accesso siano maggiormente garantiste, perché io voglio scoprire cosa c'è dentro questa situazione. E voglio sapere chi ha firmato questi atti, perché, a seconda di chi ha firmato, è possibile che ci siano forti conflitti d'interesse. Il che mi è confermato dal fatto che questo nome non lo abbiamo neanche oggi.

Signora Presidente, in relazione ai quesiti posti, la società ANAS riferisce circa i lavori sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, macrolotto 3, parte 2a, compresi tra lo svincolo Laino Borgo al chilometro 153,400 e quello di Campotenese al chilometro 173,900, per una estensione di oltre venti chilometri. Tali lavori riguardano, in particolare, l'adeguamento plano-altimetrico e geometrico dell'esistente tracciato autostradale, da svolgersi in parte in sede e in parte in variante, mediante la costruzione di numerose e importanti opere d'arte: 6 gallerie e 11 viadotti, tra cui il viadotto Italia, attualmente in corso di avanzata esecuzione da parte del contraente generale affidatario. Nella programmazione iniziale i termini di apertura al traffico dell'autostrada e la certificazione di fine lavori erano fissati in due fasi distinte per tratte: rispettivamente a luglio 2016 per i circa cinque chilometri finali e a novembre 2017 per la restante tratta. La previsione di completamento, però, risentendo di alcune criticità registratesi nel corso dell'intervento (scavo della galleria Laria e viadotto Italia), ha comportato una revisione del programma dei lavori con traslazione a novembre 2018 del termine previsto. Per tale motivo, nel quadro generale delle valutazioni condotte, si è ravvisato il vantaggio di poter disporre dell'asse autostradale completamente libero da cantieri già dall'anno corrente, rendendo fruibile il macrolotto 3 a due corsie per senso di marcia su tutta l'estensione fin dal prossimo esodo estivo, anticipando l'apertura al traffico dell'intera nuova sede al mese di dicembre 2016. Le valutazioni hanno confermato la fattibilità tecnica di tale obiettivo per mezzo di un potenziamento dell'organizzazione di cantiere, con incremento di maestranze e mezzi atto a garantire i livelli produttivi necessari per il completamento dei lavori. l'ANAS fa presente che il costo per il riassetto organizzativo del cantiere a carico del contraente generale e indicato in una prima stima pari a circa 20 milioni di euro, a conclusione delle indagini istruttorie svolte, risulta ad oggi quantificato in circa 13,8 milioni di euro. La medesima ANAS ha inoltre evidenziato che la possibilità di rendere fruibile all'utenza l'intero macrolotto in nuova configurazione, in anticipo rispetto alla data prevista, riflette un indubbio beneficio in termini di percorrenza dell'arteria in maggior sicurezza e senza i disagi derivanti dalla presenza dei cantieri. Si potrà, inoltre, verificare un ritorno positivo anche per le realtà produttive del territorio grazie ai conseguenti ridotti tempi di trasporto e ai più fluidi collegamenti verso i poli intermodali strategici. Inoltre, la possibilità di un eventuale incremento dell'importo dei lavori, in casi particolari, era stato espressamente previsto nel capitolato speciale di appalto, allegato alle lettere di invito spedite alle ditte ai fini della procedura ristretta per l'affidamento dell'intervento in questione. l'ANAS ritiene che la gara non può ritenersi alterata né nella fase partecipativa né in quella esecutiva, poiché sin dall'inizio era stata resa nota a tutte le imprese partecipanti la possibilità che l'importo potesse potenzialmente aumentare rispetto a quello iniziale. Tutte le società, quindi, hanno avuto identica opportunità di valutare tale possibilità ai fini della formulazione dell'offerta. Il medesimo discorso è applicabile nell'attuale fase esecutiva in quanto la diversità dell'importo è riconducibile all'applicazione di una norma rientrante nelle regole di gara. L'ANAS informa altresì che si sono avuti in passato altri casi in cui si è fatto ricorso alla procedura descritta, e più precisamente in quelle situazioni che individuavano un apprezzabile interesse a completare in anticipo i lavori, considerate la rilevanza dell'arteria nel sistema infrastrutturale e trasportistico e l'entità dei flussi di traffico regionale e nazionale insistenti sull'arteria stessa. Infine, circa il progetto della Valdastico Nord, riprendo integralmente quanto ho avuto modo di riferire poc'anzi: per la società Brescia-Padova, la concessione non è stata prorogata, ma è in essere non si è quindi in presenza di una proroga alla concessione scaduta ma di attuazione di quanto espressamente previsto nella convenzione che ha tra l'altro fissato il termine della scadenza contrattuale rideterminandolo, in funzione della realizzazione della Valdastico Nord, al 31 dicembre 2026.

alla lettera che disciplinano la possibilità di pagare un supplemento nel caso in cui questi lavori vengano completati in anticipo. Manifesto anche, di passaggio, una certa

stessa data e poi, improvvisamente, si è scoperto che poteva finire un anno prima. Sono piccoli miracoli che succedono e menomale; speriamo solo che non siano costati troppo (sembra che addirittura la somma di 20 milioni sia stata ridotta). Ringrazio per il dettaglio e la puntualità della risposta.

in relazione alla concessione dell'autostrada A22 Modena-Brennero, il 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) il protocollo d'intesa per l'applicazione del modello di gestione, di cui all'articolo 17 della direttiva europea n. 23 del 2014 - sull'aggiudicazione dei contratti di concessione - concernente l'affidamento dei contratti a società a prevalente partecipazione pubblica. Per addivenire a suddetta sottoscrizione il MIT, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la realizzazione delle opere strategiche di sviluppo stradale senza soluzione di continuità, ha eseguito nel corso del tempo una valutazione sulle possibili modalità di gestione del rapporto concessorio. Nell'ambito dei contatti tra il Governo italiano e la Commissione europea nel primo semestre 2015 è stata riscontrata la possibilità di applicare il modello operativo previsto dal citato articolo 17. Tale norma prevede la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal MIT, di affidare direttamente di affidare direttamente una concessione, qualora vengano rispettati i requisiti ivi previsti e precisamente che: l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul concessionario un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi; nella compagine societaria del concessionario non vi sia alcuna partecipazione di capitali privati diretti (ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportino controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati) che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Relativamente a tale ultimo requisito, il MIT si è peraltro orientato nel senso di richiedere che i futuri concessionari siano interamente partecipati da soli soci pubblici e, in aggiunta, ha manifestato l'esigenza che le società, preposte a subentrare nei rapporti concessori vigenti, non siano ricomprese nel perimetro della pubblica amministrazione, così da risultare irrilevanti ai fini della finanza pubblica. Siffatta peculiarità è avvalorata dalla autonomia economico-finanziaria delle tratte autostradali in questione, in grado di generare un flusso di ricavi superiore ai costi di costruzione e di gestione. Lo Stato e le amministrazioni pubbliche interessate hanno, quindi, convenuto di attivare la procedura di collaborazione ai sensi dell'articolo 2 della citata direttiva 2014/23/UE, secondo il quale le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. L'attività di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche è stata regolata dal predetto protocollo d'intesa nel quale si delineano e si definiscono i punti salienti dell'affidamento della concessione; in particolare le amministrazioni pubbliche territoriali e locali socie di Autostrada del Brennero sanciscono che la tratta autostradale gestita rappresenti un'infrastruttura fondamentale per la promozione dell'economia dei territori attraversati, e che quindi vada gestita in forma diretta -avendo riguardo dello sviluppo territoriale, della gestione ambientale e dei proficui risultati gestionali ed economici conseguiti fino ad oggi - attraverso un'impresa di loro emanazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 della citata direttiva. Il protocollo prefigura successive iniziative dei soci pubblici interessati dirette a modificare le attuali configurazioni societarie sia in termini di regolazione statutaria, che in termini di compagine azionaria. Nello specifico, si definiscono l'individuazione e l'adozione delle misure da attuarsi, con i necessari strumenti normativi e amministrativi, per l'affidamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle concessioni autostradali attualmente assentite ad Autostrada del Brennero SpA a società interamente partecipate da amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti all'accordo. A conclusione della procedura di cui all'articolo 17 e secondo quanto previsto dal protocollo, dovrà essere stipulato con la società concessionaria un atto convenzionale che fissi la durata della concessione, il programma degli investimenti e le modalità di finanziamento. Da quanto riportato, emerge che con la sottoscrizione del protocollo non è stata autorizzata alcuna proroga alla concessione dell'autostrada A22.

interrogativi restano senza risposta, ma su uno sicuramente la risposta c'è stata. Nel lontano agosto del 2014 chiedevo le ragioni del ritardo delle procedure

allora nelle cose e cioè, se non c'è una nuova gara, gli attuali concessionari continuano a gestirla tranquillamente, con grande beneficio loro, dei loro dipendenti - pagati più del doppio della media della pubblica amministrazione - e di tutto quel sistema di potere che c'è intorno alla Autostrada del Brennero. L'altra ragione l'abbiamo capita per l'appunto il 14 gennaio, cioè un anno e mezzo dopo aver presentato l'interrogazione: l'intenzione era di non fare la gara, che peraltro era già stata indetta dal governo Berlusconi nel 2011 e poi era stata annullata per varie vicende. Non ho avuto risposta su quali siano i tempi nei quali saranno indette le gare per le concessioni autostradali scadute o in scadenza, anche se ho avuto assicurazione dal Ministro stesso, forse qualche settimana fa in quest'Aula, che sarebbero state fatte. Però ancora non ho ricevuto risposta su questo. Ogni giorno i gestori delle concessioni in scadenza guadagnano almeno due milioni di euro: parliamo di margine, non di incasso, un margine di guadagno che potrebbe essere ben assottigliato dal meccanismo della concorrenza che si attua attraverso le gare. gare. Ogni giorno che si ritarda sono 2 milioni in più che il contribuente, attraverso i pedaggi autostradali, conferisce a queste società. È giusto che guadagnino, ma questo guadagno potrebbe essere assottigliato a beneficio o dello Stato o dell'utente automobilista. Su questo non ho ancora ricevuto

che si intende applicare una norma europea, ma non c'è l'obbligo di applicarla: è una possibilità e non un obbligo. Resta senza risposta la mia domanda sul perché non si facciano le gare.

a qualcuno, essendo controllata da enti locali, il cui governo è facile individuare in mano a chi sia. Mi ritengo, pertanto, soddisfatto, per i punti che ho ho citato, delle risposte ottenute ma faccio notare che anche questi atti, che erano stati chiesti fin da gennaio scorso (anzi, in realtà erano stati chiesti un anno e mezzo prima), ancora non li ho benché abbia fatto richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge che dovrebbe tutelare ogni cittadino; anche la commissione per l'accesso è in ritardo nel darmi una risposta. Auspicherei

forestali*. Signora Presidente, onorevoli senatori, considerata l'analoga questione rappresentata nelle interrogazioni, ho ritenuto opportuno rispondere congiuntamente. Siamo consapevoli dell'importanza e della delicatezza del tema sollevato dagli interroganti, ma è doveroso premettere che le vigenti disposizioni internazionali ed europee afferenti la materia stabiliscono precise limitazioni alla consistenza numerica delle flotte nazionali (circuizione e palangaro) autorizzate alla pesca del tonno rosso. Infatti, la vigente raccomandazione ICCAT n. 14-04 ha ulteriormente confermato, per il triennio 2015-2017, il principio generale del congelamento delle flotte (*freezing*). In particolare, per il settore della circuizione, non è stato consentito incrementare il numero degli operatori autorizzati, rispetto a quello già operante nel precedente biennio 2013-2014. Peraltro, il regolamento n. 72 del 22 gennaio 2016 ha confermato all'Italia, per l'anno in corso, un numero massimo di 12 unità autorizzabili nel settore della circuizione e di 30 unità nel settore del palangaro. Alla luce di tali disposizioni, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ha dovuto allinearsi a dette limitazioni, pena la mancata approvazione - da parte delle competenti istituzioni europee del previsto Piano annuale di pesca e la conseguente impossibilità di avviare la campagna corrente. Ciononostante, posso assicurare agli interroganti che proseguirà l'attività del MIPAAF in sede europea volta a superare dette limitazioni e ad aumentare il numero degli operatori autorizzati. Ciò posto, mi preme evidenziare che la recente sentenza n. 1100 del 2015 del TAR Lazio ha ritenuto che l'attuale regime non violi la libera concorrenza, in quanto applicativo della normativa sovranazionale di riferimento e del principio di consequenzialità per il perseguimento dell'obiettivo prioritario della politica comune della pesca. Ciò, al fine di garantire la salvaguardia della risorsa ittica mediante un rigido processo di contenimento dello sforzo di pesca e il contemperamento tra sostenibilità ambientale e redditività imprenditoriale dell'attività di pesca con il raggiungimento, entro il 2022, del rendimento massimo sostenibile. Occorre peraltro tener presente che le legittime aspettative degli operatori non autorizzati alla cattura del tonno rosso (ivi comprese le flotte cosiddette artigianali), possono essere soddisfatte già oggi attraverso le cosiddette catture accessorie. Infatti, con la corrente campagna di pesca, oltre ad avere ottenuto un ulteriore incremento (sei tonnellate) rispetto al 2015, del contingente (quota indivisa) destinato alla loro copertura, i predetti operatori hanno beneficiato anche di un aumento del previgente limite annuale (passando dai 750 ai 900 chilogrammi all'anno per imbarcazione), ferma restando la percentuale del cinque per cento ammessa, in sede di sbarco, dal richiamato quadro normativo sovranazionale. Il Ministero continuerà, con il massimo impegno, da un lato, a tutelare la risorsa ittica, e dall'altro - come detto - a garantire accessibilità e pari condizioni agli operatori del settore della pesca.

in sé delle barche, ma di congelamento della quantità di tonnellaggio delle quote di circuizione. In Italia, nonostante le raccomandazioni ICCAT dicessero il contrario, ovvero che bisognava ridurre la quantità di quel tipo di pesca, proprio perché particolarmente violenta, si è passati da 1.370 tonnellate per la sola circuizione nel 2012 addirittura a 2.050 tonnellate previste per l'anno in corso. Ancora, è vero che la sentenza del 2015 prevede che la normativa sovranazionale di riferimento dia queste indicazioni, ma ogni anno

la Francia, in questi anni, esattamente nel 2014, nel 2015 e nel 2016, nonostante partissero da un numero di barche largamente superiori a quelle italiane (42 barche in Italia, 130 in Spagna e 200 in Francia) hanno ulteriormente aumentato le autorizzazioni di pesca, ovviamente non di circuizione, proprio perché è una pesca violenta e quindi bloccata, ma per le altre barche. Segnalo ancora che le sei tonnellate - che ovviamente sono una dimensione piuttosto minima - di cattura accessoria che sono state autorizzate, di fatto sono andate, insieme alle altre, a chi già aveva le autorizzazioni di pesca, in tal modo limitando modo limitando ulteriormente, purtroppo, la possibilità per le barche che fanno pesca accidentale senza avere l'autorizzazione di pesca di non

Apprezzo il fatto che dal Ministero arrivi un'apertura per ulteriori autorizzazioni. Segnalo che inizia ad esistere un tema ambientale, perché quando le autorizzazioni per le barche sono concentrate in quattro Regioni, e la Liguria e la Sardegna, che sono le prime Regioni a a ricevere l'entrata del tonno che arriva dall'Atlantico, non hanno una sola autorizzazione di pesca

quote di pesca artigianale, sollecitato anche al livello europeo, grazie all'approvazione, nelle raccomandazioni ICCAT di un emendamento proposto da un europarlamentare ligure, l'onorevole Briano, non ha trovato applicazione in Italia, nonostante potesse trovare applicazione Concludo con un'ultima osservazione. In Italia è stato fatto un ulteriore errore, a mio avviso, che il Ministero dovrebbe tenere in considerazione. L'aumento di quota di pesca sportiva sportiva - cosa che non è stata fatta in altri Paesi, dove, al contrario, è stata diminuita - non produce altro che un'evoluzione che indebolisce il sistema di pesca organizzato e artigianale a scapito di coloro che invece della pesca ne fanno soltanto un un *hobby*. Attenderemo comunque queste nuove aperture da parte del Ministero.

Le tre tonnare possono svolgere solo attività turistica. Ciò va anche bene, perché l'importante è aver ottenuto il risultato e non aver cancellato la storia. Mi permetto di dire che Favignana vanta una grande storia sulle tonnare e sulla pesca del tonno. però, quanto mai contraddittorio aver permesso di fare tonnara turistica in maniera assolutamente sostenibile (niente di violento)

Ritengo che non sia neanche così complicato impegnarsi per dare delle risposte a breve a un territorio e, per voler essere anche più